Onorevoli colleghi, è con grande dolore che ricordo all'Assemblea l'improvvisa e prematura scomparsa, nella notte tra venerdì e sabato, del collega, senatore Luigi Scotti. Questo pomeriggio mi recherò a Cernusco sul Naviglio, sua città natale, per partecipare ai funerali. Alle ore 18 di oggi sarà celebrata in suo suffragio una messa presso la chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza. La figura del nostro stimato ed apprezzato collega sarà solennemente ricordata all'inizio della seduta pomeridiana di domani. Desidero qui però rinnovare, a nome mio personale e dell'intera Assemblea, i sentimenti da me già espressi del più profondo cordoglio e della più sentita partecipazione al dolore della famiglia, del Gruppo parlamentare del Popolo della Libertà e dei suoi elettori. Invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e l'approfondito dibattito nelle Commissioni, approda all'Aula il disegno di legge di proposta governativa n. 1209 relativo alla legge finanziaria 2009. Chi a distanza di un solo anno rispetto alla precedente finanziaria volesse stabilire dei paralleli tra l'attuale situazione e quella in cui è maturata la corrispondente norma del 2008 avrebbe certamente qualche difficoltà. Infatti, la principale novità dell'attuale disegno di legge non è nel contenuto del medesimo, ma nell'*iter* che il Governo ha deciso di percorrere, consolidando un processo in più tappe per mettere in sicurezza i conti pubblici e creare le condizioni perché anche lo Stato possa fare la propria parte nell'affrontare la sfida della crisi mondiale, che ha colpito prima i mercati finanziari e ora anche l'economia reale. Non si può oggi non rimarcare come il disegno di legge n. 1209 costituisca una novità assoluta, nell'arco degli ultimi decenni, per quanto riguarda questa tipologia di provvedimento. Infatti, il dibattito politico, in modo più accentuato negli ultimi anni, ha spesso fatto emergere la necessità indifferibile di riformare la sessione di bilancio del Parlamento, per evitare che con la legge finanziaria e i provvedimenti collegati si innescasse un processo di balcanizzazione del bilancio dello Stato, con la tutela di tanti interessi categoriali, territoriali e particolari, la cui somma difficilmente corrisponde all'interesse complessivo del Paese; anzi, talvolta, è in grado di pregiudicarlo e contraddirlo. I dibattiti condotti negli anni scorsi sulla riforma della finanziaria sono andati tutti a vuoto e, puntualmente, ad ogni autunno si ripresentava il meccanismo di una finanziaria *omnibus**,* a cui ben presto non è più bastato neanche lo sfogo rappresentato dai cosiddetti collegati per evitare di assumere dimensioni enciclopediche, assolutamente ingestibili. Ingestibili sia per il Parlamento, chiamato ad un estenuante dibattito, che nella prevedibile navetta tra le due Camere comportava mesi di discussione nelle Commissioni e in Aula. Ma anche ingestibile per i cittadini, le imprese, gli operatori professionali e gli enti locali, cioè tutti quei soggetti destinatari della finanziaria, che si trovavano di fronte un provvedimento legislativo *monstre*, costituito da migliaia di commi affastellati dei più svariati argomenti, spesso con disposizioni di dubbia interpretazione o addirittura contraddittorie. Appartiene a questo metodo di lavoro la responsabilità di aver dilatato oltre ogni misura il debito dello Stato, perché nell'inseguimento degli interessi delle singole categorie e dei territori si perdeva spesso la dimensione dell'interesse pubblico generale, provocando situazioni destinate a ripercuotersi per decenni sul complesso della comunità nazionale. Confido che quella stagione della irresponsabilità sia ormai alle nostre spalle - anche se per un paio di generazioni almeno gli italiani se ne dovranno far carico - e che la finanziaria 2009 rappresenti davvero un punto di svolta e non un episodio di questo cammino di rinnovamento. Rispetto a questo stato di cose, la cui insostenibilità era stata spesso segnalata anche da esponenti del centrosinistra nel corso della precedente legislatura, il Governo ha infatti imboccato una strada completamente diversa. Nel luglio scorso, con una manovra di respiro triennale coerente con il Documento di programmazione economico-finanziaria, ha fissato i saldi finanziari di bilancio, ponendo così dei paletti molto precisi rispetto al margine di manovra della stessa legge finanziaria, legge alla quale è stato affidato il compito di tradurre in modo organico le previsioni della manovra di luglio messe a punto con il decreto-legge n. 112, perseguendo l'obiettivo del risanamento dei conti pubblici e della migliore allocazione delle risorse disponibili. A questo riguardo appare contraddittorio il rilievo, anche da parte di quanti sostenevano da tempo la necessità di riformare i meccanismi della finanziaria ritenendoli inadeguati per un Paese moderno, di aver blindato la finanziaria e di voler imporre un testo a scatola chiusa. In realtà, come è già accaduto alla Camera, e come si conferma ora al Senato, questa è la prima legge finanziaria da molti anni che non viene varata sulla base di un voto di fiducia posto sul cosiddetto maxiemendamento, come sistematicamente è avvenuto per le precedenti, e auguriamoci che non avvenga, da molto tempo a questa parte per la necessità inderogabile di fissare un termine ultimo, sia temporale che politico alle trattative tra le parti. Si è così valorizzato, non mortificato, il ruolo del Parlamento consentendo, sia nelle sedi delle Commissioni competenti per materia che in Commissione referente, di discutere ampiamente i contenuti della manovra che, come ho già detto, non è certo esaurita nel disegno di legge n. ma si articola in un complesso di provvedimenti inevitabilmente intrecciati con gli ultimi provvedimenti governativi che hanno attuato il piano anticrisi per le famiglie, i lavoratori e le imprese. Credo si possa osservare dall'esito della discussione accademica avuto sulla riforma della legge finanziaria e del suo ruolo nei rapporti tra funzione parlamentare e funzione di Governo, che ancora una volta la politica ha dimostrato di essere materia viva, cioè un insieme di accadimenti che nel tempo riescono a stabilire una prassi e a farsi carico delle esigenze e dell'interesse comune. Le riforme studiate a tavolino, elaborate con il rigore formale dei politologi, difficilmente riescono ad affermarsi, mentre invece quando si presenta l'esigenza inderogabile di dare risposte è la stessa politica ad autoriformarsi sul campo. Sono convinto che il metodo seguito quest'anno nell'elaborazione di una legge finanziaria snella, volontariamente non onnicomprensiva ma in grado di dare risposte concrete alle esigenze per cui è nata, si affermi anche per i prossimi esercizi. Si sarà così risolto, seppure per vie e modalità sperimentali, il problema dei rapporti tra esecutivo e legislativo nella materia fondamentale della programmazione finanziaria. In effetti, è proprio con i documenti di bilancio, con il Documento di programmazione economico-finanziaria e con la finanziaria, specie in avvio di legislatura, che il Governo e la maggioranza, legittimati dal risultato elettorale, indicano con chiarezza gli obiettivi e le missioni su cui impegnare l'attività della pubblica amministrazione e le relative risorse. Se ciò non fosse avvenuto, da parte della stessa opposizione, e in questo caso a ragione, si sarebbero potute lanciare accuse di incertezza o di incapacità di dare corso al programma di Governo. Non appare neppure convincente l'obiezione che l'impostazione che ha preceduto la redazione della finanziaria dovrebbe essere in qualche modo stravolta, per dare conto degli effetti della grave crisi finanziaria che ha colpito con particolare violenza il sistema economico mondiale. In realtà, tutti i presupposti di rigore, di contenimento, di razionalizzazione, di qualificazione della spesa pubblica che erano alla base del decreto-legge n. 112 del 2008 appaiono oggi a maggior ragione adeguati. In questo dobbiamo riconoscere al Governo, e in particolare al ministro dell'economia, onorevole Tremonti, di aver agito quasi con preveggenza, stabilizzando i conti dello Stato prima che la bufera sui mercati finanziari investisse e facesse tremare economie anche più solide della nostra. Che sarebbe stato dell'Italia nelle più difficili settimane di settembre ed ottobre se il nostro Paese si fosse trovato con una finanziaria ancora aperta? Invece, con la manovra di luglio, il Governo ha dato un quadro di certezze che indubbiamente ha aiutato l'intero sistema a reggere l'urto della crisi meglio che in altre Nazioni. Pur nei margini ristretti di un percorso di risanamento che impone all'Italia di valutare con maggiore rigore di altri l'eventualità di uscire dai limiti del Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, la manovra finanziaria, nel suo complesso, contiene comunque elementi di stimolo, alcuni dei quali hanno già esercitato un benefico effetto sulle famiglie e sulle imprese. Mi riferisco ad esempio al già citato decreto-legge n. 112 del 2008, quindi alla tassazione dei guadagni di congiuntura, per concorrere, unitamente ad altre risorse, alla creazione di un fondo sociale destinato alle fasce più deboli della popolazione, fondo che oggi permette di emettere la cosiddetta *social card*, la carta acquisti per pensionati e famiglie a basso reddito. Si tratta di provvedimenti che a ragione si potrebbero giudicare parziali se non fossero stati nel frattempo integrati dalle iniziative recentemente assunte dal Governo per il piano anticrisi, con un complesso di misure che ammontano a circa 80 miliardi di euro per fronteggiare le difficoltà che attendono l'economia italiana, con il rischio recessione prefigurato dalle previsioni per il 2009 ed in vista di una ripresa che dovrebbe finalmente consolidarsi nel 2010. Lo stesso dato della diminuzione dell'inflazione con una rapidità inusitata, se può essere salutato come un elemento per molti versi positivo è il segnale evidente di un riflusso dei consumi e di un pericoloso ristagno dell'economia. Una rapida contrazione del livello dei prezzi indica, secondo una figura cara agli economisti, che il cavallo non beve ed è dunque necessario proporre provvedimenti atti a ristabilire la fiducia dei consumatori e delle famiglie, oltre che a fornire le risorse per far ripartire i consumi. Ciò ha fatto il Governo in queste settimane, muovendosi nel quadro degli interventi che tutti i Paesi europei stanno destinando specificatamente ad affrontare le conseguenze della crisi economica reale: interventi volti a sostenere le fasce deboli, a ridare fiducia, a mettere i lavoratori e le imprese in condizione di superare la situazione di difficoltà senza disperdere il patrimonio di professionalità che sarà necessario per affrontare le sfide della ripresa, anch'essa piena di incognite per la riorganizzazione dei ruoli che si imporrà indubbiamente tra le diverse economie sullo scenario mondiale. Anche di questi temi, pur non compresi negli articoli e nei commi della finanziaria, si è discusso - e molto - in sede di Commissione, confermando l'attenzione e la vicinanza del Parlamento rispetto ai problemi del Paese, al di là degli schieramenti e dei ruoli che ognuno che ognuno di noi è chiamato a sostenere. È stato un dibattito a mio avviso proficuo, perché ha permesso di sviscerare le diverse alternative presenti; ha permesso di valutare se siano preferibili interventi *spot* di effetto immediato ma di durata limitata, oppure di più ampia portata ma che possono produrre risultati sul medio e lungo periodo. Le intenzioni del Governo - e indubbiamente l'auspicio che tutti noi possiamo formulare, al di là delle diverse posizioni - è che dai provvedimenti anticrisi sorgano opportunità di riforma ampia e profonda di molti meccanismi di azione del sistema pubblico. Accenno brevemente, a titolo di esempio, al sistema degli ammortizzatori sociali, per il quale l'aumento delle risorse dedicate potrebbe essere l'occasione per una profonda riforma con l'affermazione del modello dell'assegno di disoccupazione, dando completamento alla riforma Biagi; oppure al tema della razionalizzazione dell'impiego delle risorse e strutture pubbliche che diviene, in un momento di restrizione delle disponibilità, una necessità ineluttabile. Passando all'analisi dei contenuti testuali più significativi, si osserva che l'articolo 1 indica i risultati differenziali e mantiene i saldi netti da finanziare per il 2009, determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, e fissa il ricorso al mercato finanziario in 260.000 milioni di euro. Per gli anni 2010 e 2011 i valori del saldo netto sono rispettivamente 19.800 e

Il comma 4 dell'articolo 1 contiene una norma di indirizzo, che con riferimento alla diminuzione della domanda interna destina le eventuali maggiori disponibilità di finanza pubblica realizzate nel 2009 alla riduzione del carico fiscale a favore delle famiglie. L'articolo 2 del testo, che già conteneva proroghe, agevolazioni per l'agricoltura e l'autotrasporto, così come emendato dalla Camera dei deputati comporta ulteriori interventi indirizzati a far fronte alle conseguenze più pesanti in termini occupazionali della crisi economica, con lo stanziamento di 600 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali, somma destinata a crescere con i provvedimenti già assunti dal Governo con il decreto-legge n. 185. Inoltre, si definiscono interventi per il riordino del settore previdenziale e per i contratti dei dipendenti pubblici. Nello stesso articolo 2 il testo proveniente dalla Camera dei deputati contemplava alcune modifiche ai criteri per il patto di stabilità interno. La 5a Commissione permanente in sede referente ha approvato emendamenti, alcuni dei quali con il fattivo contributo dell'opposizione, che intervengono in materia di derivati, rivedendo le modalità di stipula dei contratti di finanza derivata per le Regioni e gli enti locali e prevedendo il divieto di stipula di nuovi contratti fino a regolamentazione della materia e comunque per un anno. È fatta salva la facoltà di rinegoziazione degli attuali strumenti. patto di stabilità interno, per il quale è prevista la deroga alle sanzioni per Regioni ed enti locali che investano in infrastrutture, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. istruzione, con apposito emendamento è prevista la disposizione per stabilire entro 30 giorni i criteri per il trasferimento alle Regioni di fondi per le scuole paritarie e materne. Nel bilancio è allocato uno stanziamento di 120 milioni aree svantaggiate, è stato previsto un intervento di promozione per i territori confinanti con Regioni a statuto speciale, per complessivi 71 milioni di euro nel triennio 2009-2011. maggiori entrate a favore di CONI ed UNIRE, derivanti dall'incremento del prelievo fiscale sugli apparecchi per il gioco; contributi e interventi a favore delle associazioni combattentistiche, per la città di Gorizia e per gli italiani all'estero. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi avvio a concludere non senza sottolineare che il disegno di legge n. 1209 si colloca indubbiamente nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e come tale costituisce una risposta alle esigenze del Paese, di cui si può discutere l'impostazione, non la necessità. La gravità delle sfide che si appalesano all'orizzonte richiede, a mio avviso, da parte della classe politica un'acquisizione di responsabilità,

sia di opposizione che di maggioranza, per il significativo contributo al dibattito il presidente Azzollini, il collega Saia (relatore del disegno di legge di bilancio, che ha seguìto un percorso parallelo a quello della finanziaria) e il rappresentante del Governo, Il medesimo senso di responsabilità credo possa animare questo dibattito in Aula, utilizzando lo spazio di discussione, che spesso in passato è stato limitato dalla richiesta della fiducia, come regolarmente avveniva sulle leggi finanziarie *omnibus* da parte di Esecutivi di diverso colore politico. Al Senato, questa volta, non è stata negata la facoltà di discutere e confrontarsi su una proposta concreta, su cui si possono esprimere giudizi contrapposti come è nella logica della dialettica politica, ma a cui non si può negare di aver avuto il coraggio di porre in modo fermo i problemi del Paese e le ricette, anche difficili, per affrontarli ora, dal momento che il tempo dei rinvii sembra ormai definitivamente esaurito. *(Applausi

legge n. 1210*. Onorevoli colleghi, il dibattito di questa sessione di bilancio si è contraddistinto per un ampio e articolato confronto tra Governo, maggioranza ed opposizione sulle scelte di politica economica più idonee ad affrontare la crisi finanziaria e dell'economia reale in corso. Durante l'esame dei documenti di bilancio, la Commissione europea ha presentato, il 26 novembre scorso, il Piano europeo per fronteggiare la crisi economica. Il Governo italiano ha, poi, emanato il decreto-legge n. 185 del 2008, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale. Non è questa la sede per discutere il decreto-legge ora all'esame della Camera dei deputati; tuttavia occorre sottolineare ed apprezzare la scelta di fondo operata in questa fase. Nonostante la Commissione europea abbia autorizzato i Paesi membri a utilizzare pienamente i margini di flessibilità garantiti nelle fasi negative del ciclo economico applicando le disposizioni previste dal Patto di stabilità e crescita in presenza di «circostanze straordinarie», il Governo ha prudentemente evitato di peggiorare il deficit, tenuto conto del gravoso peso del debito pubblico. È apprezzabile il confronto svolto in Commissione nel quale l'opposizione ha criticato questa scelta proponendo di procedere, di converso, ad una manovra espansiva attraverso interventi strutturali nel 2009 ed attuando, contestualmente, misure di riduzione di spese per il 2010 e 2011 al fine di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio-lungo periodo. Tenuto conto del deterioramento dell'andamento del PIL previsto in Europa, la maggioranza ed il Governo hanno scelto di mettere in campo gli strumenti necessari per dare sostegno all'economia mantenendo invariati gli obiettivi di finanza pubblica sottesi alla manovra di luglio. Scelta, quest'ultima, non condivisa dall'opposizione, ma in ogni caso ispirata al perseguimento del giusto *mix* tra rigore e sviluppo. Passando ai temi più strettamente legati al bilancio, l'esercizio 2009 rappresenta il secondo anno di applicazione della riclassificazione del bilancio per missioni e programmi. Va ricordato, infatti, che in occasione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2008 è stata effettuata una riclassificazione funzionale della spesa rispetto al precedente bilancio classificato, invece, in chiave amministrativa. La riclassificazione è stata richiesta dal Parlamento ed effettuata dal Governo, con l'ottica di agevolare la lettura del bilancio. Cosa si intende per migliore lettura del bilancio? Negli ultimi anni, a causa della pressione del vincolo europeo unitamente all'esigenza di ridurre la pressione fiscale per sostenere la crescita e la competitività del Paese, si è manifestata l'esigenza di garantire un migliore uso delle risorse per consentire l'ulteriore consolidamento dei conti in un quadro di «qualità dell'intervento pubblico». In tal senso, lo strumento del bilancio non dovrebbe soltanto esplicitare le priorità della spesa nei singoli comparti, ma dovrebbe anche consentire una lettura dei risultati in termini di livelli di offerta di beni pubblici. A tal fine, accanto alla modifica della struttura del bilancio, sono stati ricercati spazi di manovra aggiuntiva attraverso la «revisione della spesa». Rispetto, quindi, agli obiettivi di operare scelte allocative e di disporre anche di un bilancio delle *performance* delle pubbliche amministrazioni, è possibile fare una prima valutazione dell'apporto offerto dalla riclassificazione del bilancio. La riclassificazione funzionale rappresenta, infatti, uno strumento, ed in quanto tale, è suscettibile di essere sottoposto a verifica. Forse, un anno è un orizzonte troppo ristretto per fare bilanci sugli esiti della nuova classificazione; tuttavia, è possibile trarre alcune preliminari conclusioni da questa esperienza. A ciò si aggiunga che tale valutazione deve essere esperita tenendo conto che sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ha inciso in maniera sostanziale la disciplina introdotta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. L'anticipazione della manovra triennale a luglio rappresenta un significativo elemento di novità, dal punto di vista istituzionale. Il processo di programmazione economico-finanziaria è stato dunque anticipato nella tempistica ed impostato su base triennale, al fine di conferire alle amministrazioni maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programmi di spesa di propria competenza. Gli effetti del decreto-legge, approvato prima della presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, risultano pertanto già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011. La proiezione triennale delle misure adottate avvicina il saldo di ciascuno degli esercizi successivi all'obiettivo programmatico fissato per l'esercizio, nell'ambito della programmazione di medio periodo. Solitamente, peraltro, gli effetti finanziari delle misure adottate nelle precedenti manovre non colmavano l'intera differenza tra andamenti tendenziali e valori programmatici negli anni successivi al primo. Per tali esercizi la correzione necessaria a realizzare gli obiettivi programmatici veniva, pertanto, rinviata alle manovre successive. Tale aspetto comportava una incompletezza informativa sulla composizione di medio periodo della scelta di politica fiscale, derivandone la difficoltà di valutare compiutamente la sostenibilità della programmazione di medio periodo. Se quindi in passato la correzione dei saldi era rimessa alla legge finanziaria, questo bilancio incorpora già gli effetti della manovra di luglio. Inoltre, gli interventi dello scorso luglio hanno definito le grandezze complessive, lasciando aperta un'ampia componente di scelta allocativa, da attuare in una fase successiva. Infatti, le consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie per il triennio 2009-2011 operate dall'articolo 60, comma 1, erano indicate per missioni di spesa (con evidenziazione separata della quota di fattore legislativo su cui avrebbero inciso), ma dovevano essere articolate per programmi e macroaggregati in occasione della predisposizione del bilancio a legislazione vigente. Ciò prefigurava un nuovo ruolo del bilancio, tanto più rilevante se si tiene conto del fatto che il citato decreto-legge introduceva, altresì, un margine di flessibilità per le amministrazioni in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente per il 2009, consentendo (in via sperimentale) di rimodulare, entro certi limiti, le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione, anche mediante modifica delle autorizzazioni legislative È quindi nel disegno di legge di bilancio che sarebbe possibile cogliere pienamente gli effetti complessivi della decisione operata in luglio ed esaminare la scelta allocativa proposta dalle amministrazioni di merito. Si tratta di aspetti che richiamano considerazioni più generali sul ruolo dell'Assemblea legislativa nella decisione di bilancio. È di tutta evidenza che, a fronte dell'attenuazione dei margini di decisione assunta dal Parlamento, in particolare nella sessione di bilancio, occorre decidere se privilegiare un'azione di controllo sull'allocazione e sull'utilizzazione delle risorse pubbliche al fine di conferire nuovo prestigio e nuove funzioni all'istituzione parlamentare. Nuovo ruolo che richiede, per coerenza e rigore, un più deciso apporto di informazioni ed elaborazioni, un rafforzamento che nel dibattito comune va sotto il nome di trasparenza. Da questa prospettiva l'esposizione nel bilancio di una sola parte degli effetti connessi con l'esercizio della flessibilità, quella riconducibile ai fattori legislativi, fornisce una visione necessaria, ma parziale. Tale considerazione sembrerebbe confermata dal fatto che la variazione complessiva sugli stanziamenti di bilancio riconducibile alla flessibilità sui fattori legislativi non è compensata al suo interno, ma evidenzia un risparmio di spesa, cui verosimilmente dovrebbe corrispondere una maggiore spesa assegnata sui capitoli discrezionali. il bilancio la legislazione vigente una volta che è intervenuta una manovra a luglio richiede di conoscere l'effetto delle innovazioni legislative ripartite per missioni e programmi. Ciò ha suggerito di integrare la documentazione predisposta per la sessione di bilancio con un'analisi approfondita del disegno di legge di bilancio, svolta dal Servizio del bilancio, attraverso la costruzione di un *database* in grado di raccogliere e classificare le informazioni di base delle spese per missioni e programmi a partire dal 2008,

Si tratta di un lavoro di documentazione a supporto della decisione di bilancio molto apprezzabile che, per la prima volta, mette a disposizione dei senatori un corredo di elaborazioni esaustivo del tutto inedito. Ovviamente, questa banca dati richiede di essere aggiornata nel corso del tempo attraverso un investimento in risorse umane e in conoscenze capaci di valorizzare e sviluppare ulteriormente le analisi a supporto delle decisioni. Questi sono gli strumenti di cui ci dobbiamo dotare se vogliamo perseguire con coerenza uno sviluppo della funzione parlamentare in chiave di controllo. Rispetto a questi obiettivi si misurerà la volontà e la capacità del Parlamento di adeguarsi ai tempi della democrazia. La tabella 1.1, riportata nel *dossier* del Servizio del bilancio, frutto del lavoro suddetto, riepiloga gli effetti in termini di entrate e spese e di saldo netto da finanziare (il deficit del bilancio dello Stato) da attuare con la decisione di bilancio. Il saldo a legislazione vigente passa da 50,6 miliardi di euro nel 2008 a circa 33,5 miliardi nel 2009. Tuttavia, non essendo disponibili le informazioni relative all'effetto delle norme contenute nell'articolato del decreto-legge n. 112 del 2008 suddivise per missioni e programmi (informazione mancante anche per le leggi di spesa), non è possibile ricostruire gli ambiti della decisione parlamentare di bilancio in termini funzionali. Quindi, si può innanzi tutto concludere che la sperimentazione della flessibilità di bilancio, non accompagnata da un'esaustiva base informativa che consenta di valutarne gli effetti in termini di riallocazione di risorse e di indicatori di *performance*, può rappresentare un limite alla possibilità di ricostruire i confini della decisione di spesa operata con il bilancio. La classificazione funzionale può dare il senso della scelta allocativa effettuata dal bilancio soltanto se si riesce a ricostruire la legislazione vigente per missioni e programmi. La procedura relativa all'analisi degli effetti finanziari delle leggi in corso d'anno non é ancora raccordata con la riclassificazione delle spese per missioni e programmi e ciò riduce notevolmente la lettura del bilancio in senso allocativo. L'anno passato il bilancio - per la prima volta - ha presentato una classificazione della spesa per missioni. In sostanza, è stato possibile avere uno sguardo d'insieme sulla ripartizione del totale della spesa tra le principali finalità dell'azione pubblica, indicazione che è possibile, ovviamente, ottenere anche per l'anno in corso. Ma qual è il senso di tale informazione in relazione alla decisione che viene adottata dal Parlamento con il disegno di legge di bilancio? Occorre riconoscere che con tale strumento i margini di decisione sono molto limitati. Il nostro sistema di contabilità di Stato, basato su due strumenti quali il bilancio - legge formale - e le leggi sostanziali di spesa, non consente al disegno di legge di bilancio di mettere in discussione di anno in anno tutte le spese. La decisione parlamentare si muove in uno spazio limitato tra la legislazione vigente e le spese obbligatorie e vincolate. È possibile comunque calcolare questa componente per il 2009? In termini di missioni di spesa, come già spiegato, ciò non è possibile. Un'ulteriore considerazione, più connessa al processo di gestione delle missioni e dei programmi, emerge dalla nota del Servizio del bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce 20 missioni sulle 34 esistenti. Inoltre, a ciascun programma dovrebbe di norma partecipare un solo Ministero, mentre nella struttura del bilancio per il 2009 si rilevano 11 programmi interministeriali. Occorre quindi ripensare l'attuale distribuzione delle missioni al fine di evitare sia un'eccessiva concentrazione di competenze, sia una deresponsabilizzazione dei centri di spesa. Inoltre, occorre tendenzialmente assicurare una coincidenza tra programmi e Ministeri, proprio al fine di valorizzare il percorso di responsabilizzazione dei singoli Dicasteri ed anche al fine di attribuire, in modo univoco, i risultati positivi della gestione, sia in termini di spesa che di risultati «fisici». Dal punto di vista del bilancio delle *performance* delle pubbliche amministrazioni, la riclassificazione rappresenta soltanto un primo passo. L'elaborazione di indicatori di *performance* consente poi di verificare l'efficacia e l'efficienza della spesa. Da questo punto di vista, occorre registrare un ritardo nella presentazione delle Relazioni sullo stato e l'efficacia della spesa, che avrebbero dovuto soddisfare le esigenze conoscitive del Parlamento in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di flessibilità di bilancio, di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. Ancora non appare sviluppato un *set* di indicatori che consentano al Parlamento di valutare l'efficacia e l'efficienza della spesa mentre si discute il bilancio, escludendo la possibilità di operare scelte allocative per favorire l'efficienza. Le previsioni di entrata del bilancio dello Stato esposte per il 2009 e per i due esercizi successivi nel disegno di legge di bilancio si basano sul quadro macroeconomico indicato nella Relazione previsionale e programmatica, presentata a settembre. Le previsioni di entrata fanno, quindi, riferimento ad un quadro macroeconomico antecedente agli sviluppi negativi della crisi finanziaria internazionale. Le previsioni più recenti dei principali organismi delineano un quadro più negativo per l'economia italiana e mondiale rispetto a quello disponibile in settembre.

Sarebbe pertanto opportuno disporre di una previsione aggiornata delle entrate, alla luce delle nuove informazioni e delle nuove stime sulla crescita anche se, dato il contesto attuale dell'economia globale e l'alta volatilità dei mercati, sarebbe complesso definire previsioni macroeconomiche affidabili. Una volta superata questa fase della crisi finanziaria, si potrà finalmente definire un quadro congiunturale più stabile e meno condizionato dall'attuale variabilità. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 463.904 milioni di euro e spese finali per 497.400 milioni (i dati sono riportati nella tabella 1.1). Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, sempre in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, è pari, in termini negativi, a 33.496 milioni di euro. Rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2008, l'importo del saldo netto da finanziare registra una forte riduzione, pari a circa 17 miliardi di euro, derivante da una riduzione delle spese finali pari a 12.358 milioni di euro e da un aumento delle entrate finali pari a 4.769 milioni di euro. Riguardo alle spese finali, la riduzione è quasi interamente imputabile al forte decremento delle spese in conto capitale, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2008, una riduzione di circa 14 miliardi di euro, a fronte di un aumento della spesa corrente di 1.859 milioni di euro. L'andamento della spesa corrente deriva da una riduzione della spesa per interessi (pari a 4.114 milioni e legata alla variazione degli interessi sui buoni postali fruttiferi, diminuiti di oltre 7 miliardi a fronte di una crescita, al netto di tale partita, degli interessi passivi di circa 3 miliardi) compensativa di un aumento della spesa corrente primaria di circa 6 miliardi di euro. Dall'analisi delle variazioni percentuali per missioni negli anni 2008-2011, svolta dal Servizio del bilancio e risultante dal disegno di legge di bilancio, emerge che nel complesso la spesa in conto capitale nel 2009 sarà ridotta, rispetto all'anno precedente, del 19,5 La spesa corrente aumenterà del 4,9 per cento. Negli anni successivi, il tasso di crescita della spesa corrente è pari all'1 per cento annuo, mentre la spesa in conto capitale continua a ridursi del 20 per cento nel 2010 Si registrano notevoli riduzioni della spesa per le seguenti missioni: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (meno 68,8 per cento nel 2009 per la spesa in conto capitale considerando tuttavia che parte della variazione è dovuta al venir meno dell'importo *una tantum* di 9 miliardi di euro presente sul bilancio 2008 per il ripiano dei disavanzi sanitari); agricoltura e politiche agroalimentari (circa il 24 per cento di parte corrente e 42,9 per la spesa in conto capitale per il 2009); istruzione scolastica (in conto capitale per il triennio con particolare attenzione al 2010 dove la riduzione è pari all'82,5 per cento); politiche del lavoro (meno 57 per cento nel 2010 per la spesa in conto capitale); politiche economico-finanziarie e di bilancio (meno 95,6 per cento di spesa in conto capitale per il 2010). A tali dati si affiancano le percentuali di crescita delle infrastrutture pubbliche nel 2010 e gli interventi per lo sviluppo ed il riequilibrio territoriale. Per la missione della difesa si registra una riduzione marginale della spesa corrente nel 2010 e 2011 ed un aumento significativo nel 2010 della spesa in conto capitale pari al 13 Analogamente accade per la spesa corrente della missione relativa all'ordine pubblico sebbene si registri una riduzione del 25 per cento della spesa in conto capitale nel 2010. Questi dati forniscono, quindi, la cornice di una strategia più generale di ricomposizione e di riorganizzazione della spesa. Occorre riconoscere che si tratta di numeri che riflettono una fase difficile per il Paese, impegnato in un processo di consolidamento dei conti pubblici reso ancora più arduo dalla congiuntura sfavorevole e dal gravame del debito pregresso, ma che ci pone una sfida ambiziosa, quella di giungere al pareggio di bilancio, e che ci chiede di esercitare la nostra azione per l'utilizzo più efficiente delle risorse disponibili. Veniamo alle modifiche apportate in Commissione. Gli emendamenti approvati non recano modifiche sostanziali agli stanziamenti previsti, limitandosi spesso ad apportare mere correzioni di errori materiali. Si distinguono da questa categoria l'emendamento che ha accolto una specifica richiesta della Presidenza della Repubblica, finalizzata alla riduzione delle risorse finanziarie destinate a tale organo costituzionale, nonché il finanziamento di interventi in materia di istruzione. Quest'ultima modifica è strettamente correlata a quella apportata al disegno di legge finanziaria che prevede la distribuzione delle risorse finanziarie alle Regioni con decreto del Ministro della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con quello per i rapporti con le Regioni. Il bilancio dello Stato, nell'ambito della contabilità pubblica, raccoglie gli stati di previsione delle entrate e delle spese relativi a tutti i Ministeri. Tra le spese figurano i trasferimenti agli altri organi dello Stato aventi autonomia contabile e finanziaria appartenenti al settore delle amministrazioni centrali, ossia ad organi amministrativi dello Stato e ad enti centrali la cui competenza si estende normalmente alla totalità del territorio nazionale. Nel bilancio dello Stato, ad esempio, non rientrano i bilanci delle amministrazioni locali e degli enti di previdenza ed assistenza sociale. Quanto pesa questo settore, l'unico sotto il diretto controllo del Parlamento, sul totale del deficit delle pubbliche amministrazioni? Da un punto di vista meramente contabile, utilizzando gli ultimi dati ISTAT per la notifica dell'indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il Trattato di Maastricht, il peso delle amministrazioni centrali (aggregato più ampio di quello del bilancio dello Stato) sembrerebbe essere pari all'87 per cento del deficit complessivo di tutte le pubbliche amministrazioni. Tuttavia, quota parte delle spese che sono poste a carico del bilancio dello Stato non sono propriamente oggetto della decisione di bilancio. Si fa riferimento agli interessi sul debito che, in termini di decisione di spesa, rappresentano una componente esogena determinata dai tassi di interesse vigenti sul mercato e dallo *stock* di debito. Analogamente i trasferimenti agli altri enti pubblici non rappresentano propriamente spese finali ma riflettono il finanziamento di amministrazioni territoriali cui l'attuale sistema costituzionale riconosce ambiti di competenza esclusiva. Sarebbe opportuno che il bilancio esplicitasse questo tipo di analisi anche con riferimento alla spesa previdenziale per consentire al Parlamento di verificare meglio la coerenza delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio dello Stato. Quindi, rielaborando i dati ISTAT del conto dello Stato al fine di escludere gli interessi sul debito ed i trasferimenti ad altri enti pubblici, il quadro cambia completamente, come indicato nella tabella 2 allegata. Si evidenzia che le uscite correnti del conto dello Stato conto dello Stato rappresentano circa il 25 per cento del totale delle uscite correnti delle pubbliche amministrazioni mentre le uscite in conto capitale dello Stato sono pari al 37,17 per cento delle uscite in conto capitale complessive. Dal lato delle entrate il conto dello Stato assorbe il 53,30 per cento delle entrate correnti complessive e solo il 7 per cento di quelle in conto capitale. Le restanti spese ed entrate sono afferenti agli altri enti pubblici, alle Regioni, alle autonomie locali, alle università ed agli enti di previdenza. In conclusione, il bilancio per l'anno 2009 per certi versi si distingue dai precedenti e non solo per la riclassificazione del bilancio. Da questa prospettiva, il decreto-legge n. 112 del 2008 ha costituito una novità assoluta sotto due aspetti. L'anticipazione della manovra triennale a luglio ha attribuito al bilancio il compito di recepirne gli effetti sin dall'inizio

funzionale, distintamente gli effetti della manovra di luglio da quella operata durante la sessione di settembre-dicembre. Ciò ha quindi inficiato le potenzialità esplicative della classificazione funzionale del bilancio. Inoltre, poco o nulla dell'efficacia e dell'efficienza della spesa è possibile desumere dai dati presentati in bilancio. È noto che l'elaborazione di indicatori di *performance* rappresenta un processo che può essere organicamente svolto nell'ambito di un intervallo di tempo medio-lungo (la Francia ha impiegato 5 anni ad attuare la riforma della legge organica del bilancio), tuttavia è altrettanto vero che è proprio questo processo ad arricchire di significato la stessa riclassificazione funzionale del bilancio. La riclassifìcazione, isolata da una prospettiva di più ampio respiro, finirebbe per costituire una mera operazione contabile del vecchio bilancio.

uno spossessamento del Parlamento - ho testimonianza diretta dell'inerzia con cui il Parlamento ha trattato l'argomento della revisione delle procedure di bilancio

pulsioni del Parlamento venivano canalizzate nella legge finanziaria - e ciò richiedeva da parte dei Governi la capacità di mantenere una ferma determinazione in occasione della sessione di bilancio - oggi quelle pulsioni si sono

della politica economica all'interno della loro sede naturale: la discussione sulla legge di bilancio e sulla legge finanziaria. È alquanto paradossale che, mentre nel resto del mondo si discute di come affrontare la situazione di particolare gravità che si è determinata negli ultimi mesi, il Senato esca dalla discussione sulla legge finanziaria con un mero spostamento di fondi a favore delle associazioni combattentistiche e delle scuole parificate. Per maggiore chiarezza, dal punto di vista sociale sono beneficiari molto significativi, ma non so quanto proporzionati alla gravità del momento che si sta vivendo. Se vogliamo riportare la questione nei suoi termini naturali - e cioè come strutturiamo in questa fase la politica economica -, credo che gli argomenti debbano essere essenzialmente due. Il primo riguarda il perno della politica economica che è costituito dal rigore e dalla disciplina di bilancio. bilancio. Penso proprio - me lo auguro vivamente - che nessuno all'interno di questa Aula in questo momento metta in dubbio la necessità che la politica di bilancio segua una linea di stretto rigore e stretta disciplina. Lo dico perché penso e sono convinto che ogni azione del Ministro dell'economia in questo momento debba essere guidata dal pensiero e dall'evoluzione dello *spread* rispetto ai *bund* tedeschi. Lo dico perché penso e credo che ogni pensiero del Governo debba essere dedicato al fatto che l'anno prossimo andrà in scadenza una quantità considerevole di titoli del debito pubblico italiano e che questo accadrà in un contesto di mercati finanziari in cui la concorrenza sarà molto più serrata di quanto non lo sia stata in passato. Credo, quindi, che l'obiettivo di fondo sia,

devono essere accompagnate da un'assoluta credibilità, altrimenti possono addirittura rivelarsi controproducenti. Cosa voglio dire in questo senso? Basta guardare quello che è successo al decreto n. 185 del 2008 nelle ultime settimane. Ho la netta sensazione, leggendo i giornali, che il volume di risorse fresche coinvolto dal decreto-legge n. 185 sia andato lievitando nel corso delle ultime settimane. Non riteniamo noi, non ritenete voi o il Governo che questo sia un segnale non particolarmente positivo positivo che lanciamo al mercato? Non riteniamo noi che, in realtà, la lievitazione del decreto dal punto di vista delle risorse fresche coinvolte implichi semplicemente che il Governo si rende perfettamente conto che la situazione economica e sociale si va seriamente aggravando e che lo farà ancora di più in futuro? Non pensate che i mercati non possano immaginare che domani non sarà più possibile trovare sempre e comunque la copertura a fronte di un intervento più massiccio, ma che lo si dovrà fare diversamente? Sappiamo che una politica di rigore e disciplina deve - lo sottolineo - essere credibile. Non so quanto sia credibile la strada che stiamo imboccando oggi a fronte - ripeto - di una situazione economica che nei mesi prossimi probabilmente

se si passa dalla norma che esamineremo in questi giorni circa l'estensione degli ammortizzatori sociali alle voci, per il momento, di ulteriore estensione degli ammortizzatori sociali - poi vedremo come -, non si sta dando in realtà il segnale che la direzione del rigore e della disciplina potrebbe essere seriamente intaccata semplicemente perché non ce la faremo? In questo caso il messaggio iniziale di rigore e disciplina potrebbe avere effetti controproducenti. Tutti ci auguriamo che così non sia, ma credo che a questo punto debba essere tenuto in massimo conto dal Governo. Guardate, colleghi, che se le cose stanno così è meglio fare come molti altri Governi hanno fatto, riconoscendo la serietà e la gravità del problema e affrontandolo di conseguenza.

abbia opinioni che vanno in tal senso perché andrebbero a detrimento del futuro del Paese e soprattutto delle generazioni più giovani di questo Paese.

presentati dall'opposizione - un piano che definisca con chiarezza la stabilità degli obiettivi della politica di bilancio per gli anni a venire, e che al tempo stesso tenga in dovuto conto il fatto che quando si vuole andare a coprire dal lato della spesa spesa interventi presumibilmente di carattere fiscale poi si deve anche tenere conto del fatto che i primi mordono solo in tempi non esattamente immediati.

anche di straordinaria opportunità, perché sono quelli in cui sono possibili quei cambiamenti che altrimenti sarebbero molto difficoltosi. L'esempio che trovo più interessante da questo punto di vista è il piano americano piano americano che non si limita solo ed esclusivamente al cemento delle infrastrutture ma, nel momento in cui pone l'attenzione alla questione delle energie rinnovabili, sta facendo una scelta per il dopo crisi solo per il durante la crisi. Non è solo e semplicemente una scelta di sostegno dell'economia in questo momento; è soprattutto una scelta per essere pronti ad affrontare il mondo che verrà.

la scelta di fondo di accentrare e concentrare è una scelta che in sé è difficile non condividere, se riferita in particolare all'utilizzo dei fondi europei. europei. Se c'è un problema che abbiamo avuto con i fondi europei negli ultimi anni è esattamente l'opposto: la mancanza di concentrazione e di visione per interventi che spesso e volentieri sono, per così dire, sovraregionali, che quindi non possono essere pensati a livello locale. però domandarsi naturalmente se la sola indicazione di alcuni obiettivi consenta poi che questi diventino concreti nei tempi impostici dalla situazione.

si tratta di usare risorse che erano state destinate a fini infrastrutturali, rispettando il vincolo di destinazione geografico, che, per esempio, nel fondo FAS è previsto, allora è nient'altro che una modalità di rendere più efficiente la spesa; in questo senso è certamente commendevole. Tuttavia, facciamo attenzione, perché se poi il vincolo di destinazione geografico non viene rispettato o se non rispettiamo la sostanza degli interventi che con quei fondi devono essere finanziati, allora stiamo facendo un'operazione molto diversa. Ad esempio, dal punto di vista delle politiche sociali che cosa stiamo pensando di fare che ci permetta dopo di uscirne più forti? La *social card* l'avremo sempre? Pensiamo che sia quella la nostra modalità di intervento nei confronti delle situazioni di disagio economico estremo? Sarà quella l'impostazione o, invece, sarà un altro intervento che riteniamo debba arrivare in questa fase di difficoltà? E se pensiamo ad un intervento temporaneo, non abbiamo memoria di quante volte interventi temporanei a carattere sociale che poi si sono rivelati permanenti? E quale è il costo, sotto il profilo amministrativo, di quell'intervento rispetto ad altre modalità di realizzazione? Se c'è una cosa che caratterizza il nostro sistema sociale è che i costi amministrativi che vi sono connessi sono, spesso e volentieri, addirittura superiori all'entità del beneficio per il beneficiario. Qual è qui il rapporto costi-costi benefici di quella misura? E - ripeto - in che senso costituisce un tassello dello Stato sociale che andiamo a disegnare?

Continuate ad immaginare un sistema di ammortizzatori sociali in cui la regola è la deroga e non viceversa? Se così fosse, ci ritroveremmo alla fine appesantiti appesantiti da un'istituzione sociale quale è il nostro *welfare* sempre più incapace di rispondere alle necessità future. Se si future. Se si volesse e se si fosse voluto affrontare il problema sul serio, questa era l'occasione vera per riformare il sistema degli ammortizzatori sociali.

però, come spesso e volentieri abbiamo detto, non impossibile da fare. Essa richiede un coraggio, una visione e una capacità di dare un'impostazione politica alla propria azione che probabilmente in questo caso è mancata. Potrei fare un secondo esempio,

si è avuto un rapidissimo ripensamento. È l'impostazione di fondo che critico perché segnala, ancora una volta, un problema che non vogliamo affrontare. O i crediti d'imposta sono un elemento strutturale del nostro sistema fiscale o non lo sono. Se pensiamo che siano puramente e semplicemente degli incentivi, allora la strada che il Governo ha scelto è corretta, ma se pensiamo, invece, che siano degli elementi strutturali del nostro sistema fiscale allora stiamo ripetendo, per ormai la

Ebbene, se pensate di affrontare il tema della cosiddetta fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno attraverso i crediti d'imposta dovrete risolvere questo nodo.

- questioni che la crisi stessa ci ha posto dinanzi e alle quali avremmo dovuto dare - credo - risposte in grado di metterci nelle condizioni migliori di affrontare il dopo.

rimarremo inchiodati a quei tassi di crescita e allora ricorderemo che oggi avremmo avuto la possibilità di mettere in campo quelle misure necessarie ad affrontare meglio il dopo crisi e purtroppo non l'abbiamo fatto.

quello che vediamo nella finanziaria e al di fuori di essa ha elementi di debolezza che ci preoccupano non per noi, ma per il Paese stesso.

Nei giorni scorsi, all'età di 69 anni, è scomparso Vito Gnutti, deputato nel 1992, ministro dell'industria nel 1994 con il I Governo Berlusconi e senatore dal 1996 al 2001. Rinnovo alla famiglia e ai suoi elettori i sentimenti del nostro cordoglio e della nostra umana vicinanza. Invito i colleghi ad un minuto di raccoglimento.

la crisi sta letteralmente sconvolgendo il mondo. Cambiano i rapporti tra i diversi protagonisti della competizione globale. Vengono rapidissimamente messi in discussione ruoli, ad esempio le famiglie degli Stati Uniti come consumatori globali a debito, che ci eravamo abituati a considerare stabili malgrado fosse evidente la loro insostenibilità di lungo periodo. sull'occupazione e sui redditi sono già pesantissimi, anche nel nostro Paese. Negli ultimi mesi di questo 2008 pagheremo, colleghi, un prezzo, in termini di distruzione di posti di lavoro nel nostro sistema economico, più alto - ormai è chiaro - di quello pagato nell'ultima grave recessione che abbiamo vissuto, quella del 1992-1993, che distrusse, lo voglio ricordare, più di un milione di posti di lavoro nel nostro Paese. Gli ordinativi delle imprese di settori cruciali della nostra economia, del nostro apparato produttivo, dal tessile di alta gamma fino alla siderurgia del tondino, sono già crollati del 30 In altri settori le cose vanno meglio, per fortuna, ma le aspettative sono gravemente cadute e il livello di fiducia tra gli operatori finanziari e del credito resta bassissimo. Certo, la crisi produce i fattori potenziali del suo superamento: il crollo del prezzo delle materie prime, *in**primis* di quelle energetiche, sembra aprire una stagione, ad esempio, relativamente lunga di prezzi bassi e di inflazione quasi nulla o, addirittura, negativa (anche se quest'ultimo dato non so se ce lo dobbiamo augurare). Tra i prezzi che calano c'è anche quello del denaro, anche se, almeno nell'immediato, il credito resta scarso a causa della crisi del credito interbancario. Ma questo è il punto, signori del Governo e della maggioranza: si può ragionevolmente sostenere che questi anticorpi endogeni, che nascono cioè dentro la crisi stessa e il suo manifestarsi, basteranno per avviare prima e accelerare dopo il superamento della recessione, dopo aver impedito che essa diventi depressione?

e si rimetterebbe poi, dopo la risposta affermativa, ad aspettare in attesa che gli anticorpi naturali che nascono dentro la crisi agiscano. Infatti, tutti i Governi del mondo si stanno orientando, e si sono già orientati, anche cambiando l'orientamento della politica fiscale e di bilancio che avevano deciso durante la stagione estiva, ad usare la politica fiscale e di bilancio in funzione anticiclica. Tutti i Governi del mondo meno uno, il Governo italiano, che insiste da due mesi sul sul *refrain*: la manovra di luglio non si tocca; tutto quello che c'era da decidere in termini di politica di bilancio è stato già deciso a luglio.

è il nucleo essenziale delle ragioni di contrasto tra il Partito Democratico e il Governo di centrodestra sul tema della politica fiscale e di bilancio. Nel confuso dibattito politico quotidiano si fa fatica a cogliere, ma di questo si tratta. Noi proponiamo, per il 2009, subito, una politica di bilancio di tipo espansivo che aumenti, lo diciamo chiaramente, di un punto di prodotto interno lordo il rapporto tra indebitamento e PIL per il 2009. Voi, signori del Governo, proponete una politica di bilancio duramente restrittiva. Citerò per tutti il dato: meno 19,3 per cento di spesa in conto capitale nel 2009 rispetto al 2008,

che avevate - allora meritoriamente, a mio giudizio - deciso di mettere la vostra politica di bilancio in perfetta continuità con gli impegni sottoscritti in Europa dal Governo Prodi.

e quella che proponete voi, duramente restrittiva così come definita a luglio, per giustificarsi devono rispondere ad una obiezione principale, diversa naturalmente per ciascuna di esse. dobbiamo rispondere alla seguente obiezione: come si fa ad evitare che il peggioramento determinato nel 2009 dei saldi di finanza pubblica e nel rapporto indebitamento-PIL non si trasformi in un aumento dell'onere per il servizio del debito, dato il volume globale del debito italiano e dato, naturalmente, il merito di credito del Paese? Voi, signori del Governo e della maggioranza, dovete rispondere con precisione a questa domanda: come si fa ad evitare che la politica di bilancio restrittiva non uccida il malato cui viene somministrata questa cura? cura? Noi ci dedichiamo alla nostra risposta, all'obiezione fondamentale che può essere mossa credibilmente alla nostra linea, non ho ancora sentito uno sforzo serio da parte vostra per rispondere all'obiezione fondamentale che si può muovere alla vostra linea. Abbiamo bisogno di

Noi in particolare del Partito Democratico non abbiamo bisogno di essere richiamati da nessuno alle esigenze della stabilità finanziaria, ci pensiamo da soli; meno che mai pensiamo di poter essere credibilmente richiamati da quello schieramento che, nel corso di cinque anni di Governo, ha aumentato di due punti di prodotto interno lordo la spesa corrente primaria tra il 2001 e il 2006. Infatti, diciamo chiaramente che, se fossimo al Governo, faremmo esattamente questo: presenteremmo una nuova Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria, volta esplicitamente ad ottenere il necessario consenso parlamentare, attraverso la relativa risoluzione, per modificare i saldi del 2009, al fine di dare fiato a una manovra espansiva di un punto di prodotto interno lordo. Tale manovra espansiva determinerebbe un peggioramento sul dato relativo al 2009, che noi in quella Nota proporremmo di recuperare attraverso riduzioni della spesa corrente primaria da operare nel 2010, nel 2011 e negli anni successivi, confermando sostanzialmente l'obiettivo del pareggio di bilancio per il 2012-2013. Di Di fronte a questa scelta, come si possono offrire garanzie ai mercati perché non peggiorino il nostro merito di credito? Noi sappiamo infatti quale sarebbe il prezzo enorme, catastrofico per la sua pesantezza, da sopportare per il Paese se ci fosse un ulteriore peggioramento del merito di credito determinato da uno sfondamento del bilancio. La risposta a noi sembra chiara, anche se molto impegnativa sul piano politico.

le misure immediatamente portate all'esame del Parlamento per la riduzione della spesa corrente primaria: la prima scelta, in assenza della seconda, naturalmente sarebbe irresponsabile; la prima scelta, sposata credibilmente con la seconda, Quali sono le scelte

molto rapidamente richiamerò le nostre scelte essenziali: in primo luogo, una riduzione della pressione fiscale IRPEF sui redditi da lavoro medio-bassi, in parte generalizzata (la quota maggiore per quanto riguarda il suo finanziamento), e in parte selettiva, rivolta esplicitamente a due obiettivi che consideriamo strategici.

sia inferiore al costo e alla pressione fiscale di un lavoratore maschio in una situazione equivalente. Il secondo obiettivo è rappresentato da una misura selettiva per la riduzione della pressione fiscale sulla quota di salario da contrattazione di secondo livello,

è indispensabile fare in questa fase per proteggere almeno una parte del mondo del lavoro dalle conseguenze più pesanti della disoccupazione provocata dalla recessione

di tipo universale che copra finalmente tutti i lavoratori, compresa quella parte crescente nel numero - che ammonta ormai a quasi tre milioni di lavoratori - che non ha un sistema adeguato di tutele. Per quanto riguarda le imprese, in generale proponiamo una misura apparentemente semplice: lo Stato si comporti con le imprese negli stessi termini con cui pretende che le imprese si comportino con lo Stato. Se deve pagare beni e servizi alle imprese, li paghi in tempi accettabili; se deve restituire un credito di imposta, paghi negli stessi tempi con cui pretende che le imprese paghino le imposte allo Stato. Si tratta di una scelta strategica volta a dare fiato immediatamente alle imprese, risolvendo un nodo di carattere generale del nostro sistema economico e produttivo, che vede il sistema dei pagamenti dello Stato in sistematico arretrato. In quest'ultimo caso, naturalmente, si tratta di risorse che già compongono il debito di cifre che determinano il volume globale del debito e, quindi, si potrebbero finanziare con misure che non Esamineremo meglio le proposte nel merito, ma il punto cruciale di discussione sulla politica economica e di bilancio che dobbiamo sviluppare in questa, infatti, è la sede giusta - riguarda il segno della politica economica. Voi volete una politica economica e confermate il segno di una politica economica restrittiva; noi vogliamo una politica espansiva per il 2009. Discutere delle singole misure senza avere sciolto questo nodo non ha alcun senso, a mio avviso, come ho cercato di dimostrare. Come ho già

prima di ogni altra considerazione ritengo necessario svolgere una premessa per aiutare a comprendere il nostro punto di vista sul provvedimento in discussione. Non ho alcun intento polemico, visto che sono sicuro che anche i colleghi della maggioranza più obiettivi possono convenire sul fatto che la scelta non solo di anticipare, ma anche di articolare la manovra finanziaria complessiva su più provvedimenti frammentati in decretazioni d'urgenza, evitando così di assumere nel disegno di legge finanziaria un'omogeneità di indirizzo politico, ha creato di fatto una situazione di inadeguatezza paradossale per il momento che si vive. E non mi riferisco soltanto al precedente istituzionale che, di fatto, ha determinato un totale svuotamento del ruolo del Parlamento e della Commissione bilancio proprio nell'esercizio di una delle loro funzioni più importanti, quale appunto l'esame del bilancio e delle previsioni finanziarie per l'anno successivo. Né mi riferisco alla rigidità volutamente conferita all'impianto della finanziaria, che ha fatto perdere l'occasione di una rivalutazione delle scelte di politica economica sin qui fatte per recuperare almeno un minimo di razionalità e di ordine nel processo decisionale, quanto piuttosto alla situazione contraddittoria per la quale andiamo a discutere nella sostanza una finanziaria che non si può toccare e che parte, tra l'altro, da dati ormai inesistenti. Si tratta, infatti, di dati basati su aggregati macroeconomici che non esistono più,

è evidente a tutti che l'esame del disegno di legge finanziaria si sta svolgendo nel pieno di una grave crisi finanziaria, in cui le famiglie italiane hanno già pagato con i loro risparmi una perdita di di consistenza per più di 305 miliardi di euro solo nell'ultimo anno, stando a quanto documentano i bollettini della Banca d'Italia. A poco servono le dichiarazioni del Governatore della Banca d'Italia che rimarca come questa crisi finanziaria si è già scaricata sull'economia reale, attivando una spirale dalla quale per il momento non si vede una via d'uscita.

Il rischio è che nei prossimi mesi potrà aumentare ancora di più il numero delle famiglie colpite dal dramma del disagio sociale per il mancato aumento del reddito reale di pensioni e stipendi, per i prezzi che continuano a crescere, per la perdita di lavoro, per la messa in cassa integrazione. La seconda considerazione è che le misure anticrisi approvate dal Consiglio dei ministri il 28 novembre scorso e non è un giudizio fazioso dato che è condiviso da molte associazioni autorevoli - sono insufficienti e poco incisive: c'è qualche risposta emergenziale per gli indigenti, poco per il ceto medio, nessuna scelta strutturale di medio periodo. La terza ed ultima considerazione è che il Governo, bontà sua, ha stabilito che la finanziaria non è la sede per affrontare questa grave situazione, una situazione in cui il Paese vive in uno stato di incertezza e di insicurezza rispetto al futuro, e che, in sostanza, non intende operare alcun intervento di politica economica che si discosti dalla linea di rientro finanziario, prevista dalla manovra anticipata di bilancio, mantenendo quindi, nonostante il terremoto finanziario ed economico, sostanzialmente inalterati gli obiettivi fissati nel DPEF.

con qualche proroga di agevolazione fiscale, qualche altra norma che non offre alcuna risposta alle esigenze primarie di crescita e di contrasto alla recessione. Allora, per evitare di far finta di discutere sul cosa e sul come, le nostre valutazioni e i nostri giudizi su questa finanziaria dovranno andare non tanto a quello che c'è, ma soprattutto e piuttosto a quello che non c'è e a quello che doveva esserci se non si fossero attivate iniziative confuse e velleitarie. L'errore della manovra economica di luglio appare oggi in tutta la sua drammaticità, se si pensa che il taglio dell'ICI ha sottratto alle casse dello Stato più di tre miliardi di euro mentre nel contempo ha escluso quattro milioni di famiglie che vivono in affitto e che non hanno il privilegio della proprietà di una casa. La tanto vituperata pressione fiscale al 43 per cento del Governo Prodi rimane tale, anzi, aumenta nel corso del quinquiennio e, tra il 2008 ed il 2009, sale del 3,5 per cento (pari a 16 miliardi di euro) ed è determinata soprattutto dall'aumento dell'IRPEF rispetto al decremento dell'IVA causato dalla riduzione dei consumi. Abbiamo un'evasione fiscale che l'ISTAT stima in 100 miliardi di euro all'anno e un sommerso pari a tre volte tanto all'anno, mentre con i provvedimenti messi in campo dal Governo che riguardano la non tracciabilità completa dei movimenti del denaro e la non obbligatorietà degli elenchi clienti‑fornitori

dopo che il Governo si era vantato di aver fatto finalmente pagare le tasse alle banche, alle assicurazioni ed ai petrolieri, che le hanno già scaricate sui cittadini, oggi si è costretti a ricapitalizzare le banche. Sono in molti a chiedersi che fine ha fatto la Banca del Mezzogiorno, di cui proprio non si sentiva, né si sente, il bisogno se prima non si riporta al centro dell'attenzione politica la questione meridionale, le risorse del FAS troppo spesso utilizzate per finalità non riconducibili ad obiettivi propri del fondo e per interventi in zone del Paese non ricadenti nelle aree sottoutilizzate. Sono in molti a chiedersi che fine ha fatto il Libro verde del Ministro Sacconi, di cui non si comprende come verrà finanziato, visto che non se ne fa più cenno in nessuno dei documenti di politica economica. Il Governo ha poi consolidato un sistema di servizi, soprattutto energetici e di mobilità, senza mercato, con tariffe, canoni, prezzi e pedaggi, con logiche di monopolio e senza qualità dei servizi, al punto che risulta quasi una presa in giro il blocco per sei mesi delle tariffe autostradali. Infine, la ciliegina sulla torta: tagli alla cieca, che assommano a 8 miliardi di euro solo nel 2009 e diventano 17 miliardi di euro nel 2010 e 30 miliardi di euro si tolgono soldi alle politiche sociali, a quelle del lavoro, allo sviluppo ed all'equilibrio territoriale, ai giovani ed all'istruzione. Tra il dato a legislazione vigente e il bilancio di previsione si registrano almeno 3 miliardi di euro in meno allo sviluppo economico,

Signor Presidente, se questi sono i provvedimenti che il Governo ha saputo e voluto mettere in campo, se il nostro giudizio dovrà essere dato a questa assenza di politiche di settore e politiche strutturali,

di chi fa fatica a vivere, allora il nostro voto a questa finanziaria che non c'è non potrà che essere convintamente e fermamente contrario.

è del tutto evidente il fatto che l'esame dei provvedimenti alla nostra attenzione non può prescindere da un'approfondita analisi degli effetti recati nella vita della nostra comunità nazionale dal decreto-legge n, 112, così come non si può ignorare l'attuale crisi economico-finanziaria che sta segnando la quotidianità dei cittadini e delle imprese del nostro Paese. Sul tavolo dell'odierno confronto parlamentare si colloca quindi a pieno titolo la proposta del Gruppo del PD per una politica fiscale e di bilancio volta ad imprimere per l'anno 2009 un segno positivo a favore dello sviluppo, prevedendo, al contempo, la necessità di misure di stabilizzazione nel medio e lungo periodo che possano portare ad un miglioramento della finanza pubblica, a partire dal 2010, negli anni successivi. D'altra parte, in queste giornate abbiamo raccolto affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze relative proprio alla preoccupante congiuntura economica. Nasce perciò la necessità di una riflessione strategica diversa rispetto alle scelte che hanno accompagnato e definito la cosiddetta manovra d'estate di cui al decreto n. In questo quadro si inserisce, a pieno titolo, la discussione sugli effetti provocati al comparto difesa e sicurezza dai tagli lineari apportati alle dotazioni finanziarie di questo settore. In realtà, questo importante e delicatissimo settore della vita del nostro Paese, è interessato da un vero e proprio processo di riforma, che avviene in maniera surrettizia, attraverso la riduzione delle risorse, senza chiamare l'insieme delle forze politiche, il Parlamento, ad un confronto di merito sulle strategie sottese alla funzione del nostro apparato militare di sicurezza. Com'è noto, il decreto n. 112 ha determinato una forte riduzione di fondi per questo comparto, mettendo a rischio per i prossimi anni la sua piena funzionalità ed operatività.

Tali riduzioni produrranno effetti negativi sui fondi destinati all'esercizio e quindi sulle attività addestrative del personale e sulla manutenzione dei mezzi. Sono state altresì ridotte del 7 per cento per l'anno 2009, e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010, le risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate, così come si sono decrementati i fondi per gli investimenti industriali afferenti a questo comparto. Le riduzioni mettono quindi in discussione tutto il quadro di alimentazione dello stesso modello di difesa. In buona sostanza, le proiezioni su base triennale 2009-2011 pongono il rischio di un progressivo decadimento operativo dello strumento militare, con una drastica diminuzione delle esercitazioni, delle ore di moto e di volo delle varie componenti, nonché una riduzione delle attività manutentive sui sistemi d'arma in inventario. Si evidenzia, ancora, il possibile insorgere di una situazione di difficoltà nel settore delle scorte operative e strategiche, nonché nella gestione dell'ammodernamento infrastrutturale. È noto poi che le restrizioni previste con il decreto citato hanno dato luogo alle proteste di tutti gli organismi rappresentativi del settore della difesa e della sicurezza. A tale proposito, ricordo che le risorse stanziate per i miglioramenti economici per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ammontano complessivamente a 586 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, corrispondenti ad una media di 67 euro mensili *pro capite*, cifra di gran lunga inferiore rispetto ai 135 euro mensili *pro capite* stanziati dal precedente Governo Prodi. Le stesse risorse - pari a 12 milioni di euro - stanziate dalla finanziaria in tabella A, così come i 60 milioni di euro previsti dal decreto n. 185 (assegnati in via sperimentale quale detrazione fiscale al personale con un reddito annuo fino a 35.000 euro), non corrispondono efficacemente alle giuste aspettative di chi è impegnato quotidianamente in attività delicatissime quali la difesa, la sicurezza e il soccorso. Risulta ormai evidente quindi, con particolare riferimento alle specifico settore delle Forze armate, che gli che gli interventi adottati dall'attuale Governo possono comportare la dissoluzione del progetto, iniziato nel 2000, relativo alla professionalizzazione del modello di difesa a 190.000 uomini, e il definitivo superamento del tradizionale schieramento lungo i confini e negli spazi territoriali nazionali. Il nostro Gruppo, comunque, non si sottrarrà assolutamente ad una discussione di merito sull'argomento, che sia in grado di contemperare le esigenze di un moderno sistema di difesa e sicurezza con i problemi connessi alla qualificazione e alla riduzione della spesa pubblica. In ogni caso è il Parlamento, in un serio e costruttivo confronto, anche su opzioni diverse, il luogo in cui verificare - credo - la validità del nostro modello di difesa, così come la possibilità di una sua eventuale razionalizzazione e riforma, e non certo, quindi, il ricorso a semplici e spesso non giustificati tagli alle dotazioni finanziarie di uno dei settori più delicati ed importanti del nostro sistema Paese. *(PdL)*. Signor Presidente, parlerò soprattutto delle ripercussioni sul bilancio della difesa

non perché faccio parte della maggioranza, ma perché era ora che si affrontasse con vera serietà la situazione finanziaria del Paese. le decisioni, naturalmente non posso fare a meno di constatare che i forti tagli che sono stati apportati alla spesa hanno avuto ripercussioni molto gravi e dure sul bilancio della difesa e si potrebbe dire che piove sul bagnato, perché il bilancio della difesa è sempre stato in situazione critica, non soltanto in termini contingenti, a seguito di quello che è accaduto nella finanziaria e legge di bilancio per il 2009, ma perché da sempre ma perché da sempre la classe politica italiana rivela, rispetto alle classi politiche dei Paesi con i quali amiamo confrontarci, una scarsa stima ed una scarsa considerazione dell'importanza del problema della difesa. Basti pensare che un cittadino italiano spende 250 euro per la difesa, mentre un cittadino tedesco ne spende 350, un

mentre abbiamo speso per la difesa la metà di quello che spendono quei Paesi. Dal momento che anche nel sociale non spendiamo più di questi tre Paesi, mi piacerebbe sapere dove vanno a finire i nostri soldi e per questo vedo con grande favore le decisioni drastiche assunte nella finanziaria. Il problema del bilancio della difesa non è un problema contingente, quindi, ma è un problema politico; è tuttavia difficile sperare che la nostra classe dirigente si decida ad uniformarsi a quello che accade normalmente nell'ambito dell'Unione europea, vista anche la grave situazione economica che sta condizionando l'operato dei Governi in tutto il mondo. È tuttavia auspicabile in un prossimo futuro che i nostri rappresentanti, che in sede internazionale sono sempre molto pronti ad assecondare le richieste di partecipazione dello strumento militare italiano alle alle importantissime e assai considerate operazioni di pace, si decidano poi anche a sostenere lo strumento, anche per evitare che si vanifichino, con una scarsa considerazione internazionale dovuta ai pochi soldi che vengono dedicati alla difesa, i sacrifici e l'impegno meritorio dei nostri soldati.

il 2009. Si possono anche auspicare, e qui mi rivolgo proprio al Governo, alcune procedure diverse per evitare certi dissesti che si manifestano in sede di Ministero della difesa

l'ipotesi finanziaria fissa alla quale possono fare riferimento nel momento in cui preparano il progetto di piano di spesa per l'anno successivo. Se non vi è questa ipotesi fissa, ogni volta accade che il Ministero fa un progetto di bilancio di spesa, naturalmente il Ministero dell'economia e delle finanze taglia regolarmente e tutto il progetto viene sconquassato. Poiché il Ministero della difesa non è un Ministero come gli altri, perché è il sostenitore di un sistema, di un progetto, di una macchina che deve continuare a funzionare a differenza di tanti altri Ministeri, è opportuno che d'ora in avanti si dica chiaramente, come in parte comunque è già stato fatto per il 2010 e per il 2011 ma deve essere fatto anche per gli anni successivi, quali sono le risorse di cui il Ministero può disporre, altrimenti la programmazione salta.

a prescindere dalla facoltà che il Ministero dell'economia e delle finanze (e comunque il Governo) ha di stabilire i limiti di spesa: questo nessuno lo mette in discussione. Entrando nel merito del bilancio per il 2009,

di chi stigmatizza l'entità delle risorse messe a disposizione le 18.000 lire per il rinnovo del contratto fissate dal Governo del 1996-2001), considerata anche la situazione economica attuale, per l'ammodernamento ed il rinnovamento pur avendo ridotto le risorse

i carburanti, le munizioni, le ore di volo dell'Aeronautica per preparare i propri piloti, la manutenzione degli aerei e degli elicotteri - sono assolutamente insufficienti. Se entro il mese di giugno o di luglio non arrivano nuove risorse la macchina si ferma: è molto semplice.

e altri 26 milioni di euro per il funzionamento. Quante volte abbiamo sentito dire, grazie anche alla stessa linea seguita dal Governo precedente, che le macchine dei carabinieri hanno

speso per le operazioni di pace, elemento fondamentale della nostra politica estera. Infine, è da apprezzare la decisione in ambito finanziario di finanziario di riconoscere l'atipicità della professione militare e delle forze di polizia. Si ringrazia per i 12 milioni di euro a messi a disposizione. Ciò rappresenta certamente uno sforzo commendevole,

quanto affermato dal Presidente della Repubblica in sede di Consiglio superiore delle Forze armate: «È ineludibile mantenere per le Forze armate capacità di intervento adeguate alle esigenze di sicurezza internazionale». *(PD)*. Signor Presidente, solitario rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, forse - anzi senza troppi "forse" - il passaggio in quest'Aula della finanziaria per che poi nel nuovo impianto di base triennale, con una folle blindatura, dovrebbe estendersi in sequenza peggiorativa anche al 2010 e 2011 - è già stato deciso e sigillato in altro tempo e in altro luogo, dove, a quanto pare, vigono la volontà e la norma di ignorare alcune delle più impellenti esigenze ed elementari aspirazioni degli italiani in Patria e all'estero. Tuttavia ciò non può costringere molti di noi a fare la parte dei ciambellani e rinunciare alla denuncia forte e circostanziata di un documento che, pur in un clima generale di crisi economica, poteva e doveva essere meglio impostato, più equilibrato e meno punitivo. Lascio ad altri colleghi, e per altri momenti quali quelli di eventuale illustrazione di emendamenti, affrontare nel dettaglio gli aspetti più gravi e l'impatto sociale, economico e politico devastante del disegno di legge n. 1209 che stiamo discutendo. Nei pochi minuti concessimi mi preme ricordare in particolare che questa finanziaria, fra l'altro, rappresenta, per le politiche per gli italiani all'estero, un immeritato colpo di una pesantezza senza precedenti. In un bilancio della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, già ridotto all'osso, di 73 milioni di euro per l'anno ancora in corso, sono stati apportati senza necessità, senza logica e senza criterio

i contributi per l'assistenza diretta e indiretta ai connazionali indigenti fuori d'Italia, che passano da 31 milioni a meno di 12 milioni l'altro scriteriato taglio di 92 milioni di euro nel bilancio della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli esteri, che contribuirà ad incidere ancora più negativamente sull'immagine dell'Italia all'estero, ci si trova di fronte allo smantellamento del sistema «italiani nel mondo», come è stato faticosamente e tanto produttivamente costruito da mezzo secolo e come lo conosciamo oggi. Mi si consenta di notare sommariamente un paio di punti. Il primo è che i tagli di 45 milioni di euro nel bilancio della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie rappresenta una cifra che è sì questione di vita o di morte per le strutture degli italiani nel mondo, ma è di tale esiguità nel contesto generale della legge finanziaria da poterla giudicare solo come espressione di una volontà politica punitiva e vendicativa nei confronti degli italiani nel mondo. Una cifra di tale esiguità recuperata, almeno parzialmente, nelle pieghe del bilancio, così come avvenne per l'ultima finanziaria, quella dell'anno ancora in corso, del precedente Governo. Il secondo punto è che il taglio di 19,5 milioni di euro nei contributi agli enti gestori dei corsi di lingua e cultura e il quasi azzeramento dei contributi per le attività culturali gestite dalle rappresentanze consolari - da 3,5 milioni a 996.000 euro - vengono a contraddire e vanificare le stesse prese di posizione ufficiali del Governo e, in particolare, del ministro Frattini circa una ripresa dell'iniziativa culturale italiana nel mondo. Ma di quale iniziativa si parla se l'Italia non ha avuto finora, e men che meno l'avrà d'ora in avanti, una coerente e coordinata politica culturale degna del nome? Se dobbiamo solo vergognarci quando le nostre politiche culturali all'estero sono messe a confronto con quelle di Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Olanda, Grecia e di un'altra ventina di Paesi di cui siamo fanalino di coda? Se la maggioranza dei corsi di italiano all'estero dovrà ora venire soppressa e le scuole dovranno letteralmente chiudere? Per il futuro dei giovani di origine italiana che in questi giorni per ironica coincidenza con la discussione della finanziaria per il 2009 si riuniscono a Roma grazie allo stanziamento di 2 milioni di euro del Governo Prodi decurtato di 600.000 euro da questo Governo Governo - c'è un vuoto assoluto di iniziativa pubblica. Non c'è più alcuna trasmissione di lingua e cultura, non c'è più politica di recupero linguistico e culturale delle seconde generazioni. di chi nella maggioranza non perde occasione di agitare il tricolore, di riempirsi la bocca di italianità, identità italiana nel mondo, italiani all'estero risorsa dell'Italia, ambasciatori di cultura, promotori del *made in Italy*, e poi in quest'Aula, come già alla Camera, non arrossisce nel votare una misura che, negando un contributo quasi insignificante nel contesto del bilancio dello Stato, distrugge i corsi di quella lingua che è ragion d'essere dell'identità culturale e della stessa presenza italiana all'estero.

preme fare una premessa, per noi importante. Abbiamo la fortuna che il ministro Tremonti e il Governo hanno deciso di anticipare a luglio la manovra. Questa è la più grossa fortuna che ci consente oggi di essere qui serenamente a discutere di legge finanziaria.

Ora, curiosamente, abbiamo sentito dire da parte di qualche esponente dell'opposizione, poco attento a quanto è stato fatto dal Governo Prodi nei due anni passati, che si poteva fare di più e meglio sul fronte del contenimento della spesa pubblica. Su questo direi proprio di no. Ho rivisto i dati, anche perché è giusto avere un minimo di memoria storica. Ebbene, la prima finanziaria Prodi entra con maggiori spese per 27 miliardi; dopo il cinema dell'assalto alla diligenza i 27 miliardi diventano 30, quindi 3 miliardi in più: alla faccia del rigore, tanto sbandierato da Padoa-Schioppa! Le maggiori entrate della prima finanziaria Prodi erano 4,4 miliardi in entrata e diventano 6 in uscita: un altro miliardo e mezzo in più di tasse. La differenza viene coperta con tagli lineari alla spesa che poi non ci sono stati, perché abbiamo dovuto rimpinguare con i cosiddetti tesoretti i tagli inesistenti.

perché era fatta di tutto e di più, i 20 miliardi diventano 24,3. Quindi 4,3 miliardi di maggiori spese nell'assalto alla diligenza,

di politica economica, di rigore nell'ambito di quanto va fatto oggi alla luce della crisi internazionale, cercando di fare il meglio possibile con le scarse risorse a disposizione. Per inciso, perché questo poi è il dato che ci mette tutti quanti in difficoltà, maggioranza e opposizione, perché siamo tutti nella stessa barca (se ogni tanto ce lo ricordiamo fa anche bene), la spesa totale dello Stato è passata da 703 miliardi prima dell'avvento di Prodi ai 780 di oggi; quindi quasi 80 miliardi di spesa pubblica in più,

(a memoria d'uomo sono rarissimi i licenziati nella pubblica amministrazione, mentre nel privato ogni giorno si rischia il posto di lavoro). Quindi, maggiore spesa maggiore spesa rigida e maggiore entrata - ahinoi! - aleatoria, perché l'anno venturo sapremo - lo sappiamo già adesso - che avremo problemi per mantenere un certo livello di entrata, in particolare alla voce IVA e non solo.

Avendo alzato l'asticella della spesa pubblica così tanto (a 780 miliardi di euro) e in così poco tempo e trattandosi soprattutto di spese rigide, quello che si può fare oggi sul lato delle entrate è davvero poco.

Combattere l'evasione fiscale significa fare qualcosa affinché, ad esempio, in Umbria non ci sia più un'evasione IRAP del 44 per cento, che non è da Paese civile.

delle cose giuste. Va bene concentrare gli interventi e gli investimenti soprattutto sull'uso delle risorse comunitarie. È una gran bella cosa: pochi interventi e pochi investimenti che si vedono. E sarebbe davvero opportuno farlo. Anche qui, però, per memoria storica

Non si riesce ad attivare un investimento di un miliardo e mezzo sulla viabilità secondaria neanche in dieci anni, figuriamoci in due, come si voleva fare! Per non dire della qualità della spesa. Il mio collega Filippi si era divertito a fare un calcolo sull'intervento previsto per la Salerno-Reggio Calabria: 11 chilometri di strada, 20 milioni di euro stanziati per la segnaletica. che, se si dipingono le strisce, vengono fuori 266.000 attraversamenti pedonali, che fisicamente non ci stanno neanche. Oppure, se si mettono semafori, viene fuori un semaforo ogni 20 metri. Questa era la qualità della spesa di certi investimenti che ancora vengono ricordati negli interventi dei nostri colleghi dell'opposizione, i quali si lamentano perché sono stati tagliati: per fortuna sono stati tagliati rami secchi come questi! questi! Concludo con la vera sfida che ci trova tutti d'accordo, ma ancora tutti poco consapevoli. L'unico modo per uscire dal tunnel è tagliare la spesa pubblica.

Per non dire delle piccole e piccole-medie imprese: uno studio dell'Associazione piccole imprese (API) di Torino arriva a stimare addirittura nel 66 per cento quanto paga una piccola impresa di tasse, la quale poi deve competere con la sua omologa spagnola che di tasse paga il 20 Questo è il problema, altro che combattere l'evasione fiscale! Qui si tratta di far sopravvivere il nostro sistema produttivo, che è fatto principalmente di piccolissime, piccole e medie imprese. Sotto questo aspetto è ottima la posizione del Governo, che ha accolto la richiesta forte e pressante della Lega di bloccare gli studi di settore e procedere ad una revisione congiunturale tenendo conto della situazione

che ogni cittadino può vedere, basta che esca di casa, soprattutto per quanto riguarda la voce «personale», che spesso è utilizzato male se non addirittura in maniera clientelare. Ebbene, se avessimo il coraggio di portare a compimento in tempi rapidi e con serietà questa grande manovra di riorganizzazione sia della spesa che delle entrate, faremmo veramente bene, una volta per tutte, a questo strano Paese. *(Applausi del

il giudizio sulla manovra finanziaria impostata mesi addietro, con un modello di tagli orizzontali, che non hanno lasciato intravedere un discernimento operativo e, quindi, progettuale per l'anno entrante e i successivi, non migliora se poniamo attenzione ai diversi decreti e disegni di legge che si stanno succedendo, con i quali il Governo intende corrispondere alla situazione di grave e preoccupante crisi della finanza e dell'economia con interventi puntuali e per settori specifici. Manca, a quanto pare, una visione d'insieme, che consenta alle cittadine e ai cittadini italiani di guardare con meno preoccupazione ai prossimi mesi. Condividiamo tutti, credo, che di fronte a così grave emergenza sarebbe utile e profittevole per il Paese un atteggiamento più positivo e, per così dire, corale da parte di maggioranza e minoranza parlamentari; occorrerebbe, tuttavia, un approccio diverso da parte del Governo verso le istanze della opposizione. In questo senso, una più marcata e sistematica azione di sostegno ai redditi delle famiglie, una precisa scelta di investimenti pubblici gestiti razionalmente e non a pioggia, una più coraggiosa azione di garanzia per le piccole e medie imprese costituirebbero segnali incoraggianti per una prima, forte risposta al preoccupante quadro che ci sta davanti. Esaminando ora molto brevemente le previsioni sul bilancio del Ministero dell'ambiente e le quattro missioni allo stesso riferibili, non può sottacersi il drastico calo di risorse riguardanti lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio. In particolare, sono stati tagliati investimenti nel contesto del programma di conservazione dell'assetto idrogeologico, con specifico riferimento agli interventi di tutela del suolo in Sicilia e Calabria e al capitolo relativo ai piani strategici nazionali; sono state drasticamente ridotte le risorse sul programma di tutela di fauna e flora e salvaguardia della biodiversità; è stato ridotto il fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra; è stata pesantemente ridotta la dotazione dei capitoli afferenti piani di disinquinamento e interventi urgenti di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. La riduzione, poi, delle risorse sulla missione relativa alla ricerca ed innovazione sembra mettere in dubbio l'avvio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), voluto dal decreto-legge n. 112 e destinato a sostituire APAT, INFS e ICRAM. Non convince - anzi, preoccupa - invece ritrovare una parte, sia pure minima, delle risorse tagliate dal bilancio del Ministero dell'ambiente, direttamente sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con destinazione a «concessione di contributi», secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 112: un modello di intervento, sostanzialmente a pioggia, secondo la tipologia della "legge mancia", che non fa prevedere nulla di buono quanto a sistematicità, coerenza ed efficacia degli interventi di risanamento e recupero ambientale e sviluppo economico, previsti come finanziabili. La recente proposta di riduzione retroattiva del beneficio fiscale per la ristrutturazione ambientale degli immobili - ora, pare, rinunciata - costituisce un segnale molto preoccupante di una complessiva disincentivazione di politiche ecovirtuose. Emblematico resta l'atteggiamento di fronte alla prospettiva 2020 dell'Unione europea in materia di obiettivi da perseguire per combattere i cambiamenti climatici in atto. La crisi economica diventa occasione, per il Governo e per Confindustria, per un drammatico ridimensionamento delle azioni prevedibili per centrare i tre «20 per cento»: di energia con fonti rinnovabili, di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni di gas serra rispetto ai 1990. Siamo, viceversa, convinti che anche la crisi economica sia una occasione propizia per interventi ed investimenti nella giusta direzione, catalizzatori di indotto importante e di prospettive di qualità. Per questo stesso motivo, in effetti, siamo altrettanto convinti che gli incentivi, anche di natura fiscale, per comportamenti e scelte individuali, familiari o collettive nel senso del miglioramento in campo energetico, ovvero per la riqualificazione, sotto questo profilo, del patrimonio immobiliare, siano non tanto da bloccare per gli anni avvenire, come purtroppo previsto, ma piuttosto da incrementare.

sviluppo: sta incardinata dentro i ritmi di crescita di una società, di un'economia e si manifesta in forme irregolari, cicliche, talvolta imprevedibili. Certe volte la connessione tra crisi e sviluppo è così accelerata, così difficile e certe volte così prolungata che qualcuno più bravo qualcuno più bravo di me potrebbe sostenere che lo sviluppo è una figura della crisi. Tuttavia, al di là del gioco nominalistico, crisi e sviluppo sono profondamente connessi, sono un binomio strutturale, un'unità ontologica che andrebbe affrontata con uno spirito dialettico progressivo. È difficile immaginare un buon destino per una politica economica che poggia, per sua dichiarata scelta, soltanto sullo slancio di misure restrittive. Bisognerebbe potere immaginare, come ha provato a fare il senatore Morando, un gioco di riscontro tra misure restrittive e misure di tipo espansivo. La maggioranza ha affrontato questa difficile situazione - che ovviamente non dipende solo dalle scelte del Governo, ma da una congiuntura internazionale particolarmente grave e di difficile soluzione

in cui sostanzialmente si annunciavano tagli orizzontali a tutto l'insieme della spesa. Questo decreto

un decreto aprioristico che ha stabilito dei lineamenti restrittivi per due o tre anni. I provvedimenti che vengono dopo sono collegati a questo in una logica smembrata e risulta perfino difficile intervenire su questo singolo provvedimento perché, in realtà, gli effetti del decreto precedente e della sua logica ridondano un po' sul

altri colleghi più esperti di me hanno affrontato i lati tecnici della questione, ma intervengo per qualche momento con alcune osservazioni critiche che possono essere fatte soprattutto in ordine alla alla logica restrittiva. Prima, però, vorrei dire una parola sulla qualità dell'espansione,

La crescita è un bene in sé? Forse, se aumentano i redditi e se aumentano le occasioni di lavoro. Però questa Però questa è proprio la circostanza messa in dubbio dal procedere di questa alternanza tra crisi e sviluppo. Grosso modo, quando c'è lo sviluppo aumentano un po' i posti di lavoro e aumentano un po' i redditi, sempre molto meno di quanto aumentano i guadagni delle imprese, i profitti e gli effetti generali di appropriazione privata delle risorse pubbliche. Quando c'è la crisi, invece, sostanzialmente i colpiti sono

dai processi della crisi, o perlomeno ci prova. Quando il sistema delle grandi imprese si trova di fronte a condizioni di inenarrabile difficoltà, esso ricorre a un espediente che è classico nella storia del capitalismo, che in Italia è conosciutissimo, che è quello - grosso modo - della socializzazione delle perdite. Prima c'è la privatizzazione degli utili e, nei momenti di difficoltà, c'è la socializzazione delle perdite, ormai teorizzata anche apertamente. Sistemi economici grandi, macro, possono tranquillamente stabilire che risanano i deficit delle banche e delle grandi imprese, cioè i deficit del deficit del mondo produttivo visto dal lato dell'intrapresa e dell'imprenditore. Nessuno pensa mai a sanare i debiti dei redditi; dei redditi; questi passano nel sacco della storia e vengono rapidamente consumati, metabolizzati e annichiliti.

di aree urbane, di dilatazione pressoché inarrestabile non solo dell'area urbana propriamente detta, ma anche di quella che gli specialisti definiscono campagna urbanizzata. È una sorta di di *sprawl* urbano (come usano dire gli urbanisti), di diffusione non a macchia d'olio, ma ramificata, tentacolare, molecolare, differenziata nello spazio, attorno ai grandi sistemi di relazione di aree, di grandi infrastrutture e così Questa espansione spesso è insensata. L'Italia rigurgita di capannoni eretti ma vuoti, di case costruite per abitazione ma non abitate; nel frattempo gli affitti urbani salgono molto più di quanto sarebbe lecito calcolare sulla base dell'offerta ipotetica di abitazioni per quelli che non ce l'hanno. C'è una strana meccanica, che qui non posso e non so risolvere; essa, però, appare abbastanza chiara agli occhi di un'analisi, anche frettolosa. Questa espansione è sbagliata, distorta e soprattutto consuma spazio, consuma la risorsa primaria; spesso consuma non solo territorio, ma anche paesaggio, mangiandolo e restituendolo avvelenato.

mangia, letteralmente, l'unica risorsa su cui potrebbe contare in una situazione difficile, dove i mercati vanno alla ricerca del lavoro a basso costo in altre zone. quadro problematico e difficile da risolvere. In tale situazione ci si aspetterebbe che un punto di vista non necessariamente progressivo, ma anche semplicemente capace di tenere conto dell'insieme delle forze affrontasse il problema del controllo sulla ripresa economica con un minimo di previsione e di capacità di incidere sui fattori dinamici e progressivi.

la manovra manca completamente l'obiettivo; anzi, non lo manca, perché non se lo pone nemmeno, è una cosa che non la riguarda. Ciò è abbastanza impressionante perché non c'è neanche l'intenzione di affrontare un argomento di questo tipo.

Il Governo precedente prevedeva per il 2009 3.862.000 euro per l'istituzione dell'Autorità per le garanzie della comunicazione

In una situazione in cui c'è chi si può permettere, tramite capitali ed autofinanziamenti, un largo, ampio ed inarrestabile possesso delle fonti di comunicazione può fare quello che gli pare, i piccoli editori ed i giornali indipendenti, che tirano la carretta a fatica e che non hanno mai i soldi sufficienti per pareggiare il bilancio, sono messi di fronte non allo spettro della riduzione ma allo spettrodella chiusura. caso particolare della democrazia italiana su cui non cesseremo mai di sollevare l'attenzione perché è uno dei più pericolosi: rinunciare alla ricerca è già terribile, ma rinunciare preventivamente alla libertà di informazione delle fonti indipendenti è un delitto.

Mi consenta, signor Presidente, in apertura una brevissima dichiarazione pubblica relativamente al mio testamento biologico. Voglio, infatti, lasciare agli atti della seduta odierna del Senato che, se mi dovessi trovare nelle condizioni di non potermi esprimere, confermo di non volere nessuna forma di accanimento terapeutico e, come tale, intendo anche l'idratazione e l'alimentazione forzata. Venendo al tema della finanziaria, è ormai noto a tutti che la manovra di bilancio che stiamo discutendo ha visto anticipati gran parte dei suoi effetti dalle disposizioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, che ha definito lo scenario finanziario per il prossimo triennio. Ed è quindi altrettanto noto che i tagli previsti nel settore della difesa hanno avuto diverse autorevoli testimonianze di allarme e di diffusa preoccupazione, non solo dalle file dell'opposizione in Senato, ma da quanti esercitano le massime responsabilità tecniche di comando nel nostro Paese. Si tratta certamente di competenze indiscusse e non ascrivibili ad alcuna parte politica, competenze che hanno segnalato nelle sedi istituzionali dovute grande preoccupazione per il rischio concreto che, con i tagli previsti, si determinino modificazioni così sensibili del sistema difesa da far temere concretamente che si produca inefficacia e inefficienza. È noto che il nostro Paese impegna per la difesa lo 0,94 per cento del PIL, mentre la Francia arriva all'1,73 per cento e la Gran Bretagna al 2,20 e comunque la media europea si assesta all'1,42. Con questo Governo, al di là dei proclami muscolari del Ministro, non siamo neanche alla storica frase dell'«armiamoci e partite», dato che la quota di risorse destinate all'Esercito risulta così ridotta negli anni da non garantire nemmeno i soldi per un numero adeguato di esercitazioni e quindi per la sicurezza diretta di uomini e mezzi, né all'estero, né tanto meno in Italia. Un esempio minimo e concreto di quanto questo Governo non abbia davvero a cuore la funzionalità del sistema, sta nel fatto che questa estate mentre si impegnavano 3.000 uomini nell'esercito nella cosiddetta operazione di sicurezza, considerata dai più di pura facciata, in realtà si tagliavano i fondi per l'ordinaria manutenzione. Ecco allora che ad agosto diverse volanti di Polizia e Carabinieri, che già usano mezzi vetusti, non sono state neanche in condizione poter fare il cambio delle ruote in dotazione per l'inverno. Solo a volersi soffermare poi sulle previsioni di contenimento della spesa sul fronte del personale, è stata indicata una modifica così significativa che trasforma sostanzialmente il modello professionale di difesa, indispensabile a far fronte alle innumerevoli mansioni oggi previste e peraltro già approvate in Parlamento, Parlamento, luogo deputato a tali decisioni. Ancora: dalle audizioni in Commissione è stato confermato che se si applicheranno i tagli previsti si tornerà a livelli inferiori al 2006, tanto da giungere al 2011 in un quadro anacronistico di insicurezza programmatica, pregiudicando l'efficienza operativa delle nostre Forze armate. Si giungerà alla riduzione dei nuovi arruolamenti ed anche al mancato trattenimento dei soldati che sono già nelle Forze armate da cinque o sei anni e che non dovrebbero che non dovrebbero vedersi congedati dopo aver prestato con merito servizio in Italia e all'estero. Non sfugge a nessuno che questi uomini e queste donne sono per la stragrande maggioranza del Sud d'Italia. Nessuno crede inoltre che tutti questi volontari del Sud e delle isole abbiano maggiore amore di Patria rispetto ai ragazzi di altre Regioni. Appare più plausibile dunque pensare che il ricorso alla leva volontaria sia anche un modo per trovare un lavoro reale in un luogo dove di lavoro se ne trova sempre meno. Seguendo tali considerazioni ho presentato con i colleghi senatori del Partito Democratico un ordine del giorno, condiviso in Commissione sia dai colleghi della maggioranza che dal rappresentante del Governo, affinché proprio il Governo assuma le misure utili a garantire la continuità del rapporto di servizio dei volontari delle Forze armate richiamati o trattenuti e che, anzi, dia attuazione alle assunzioni del personale necessario alle Forze armate e alla Polizia. Non può sfuggire onestamente a nessuno che se questa estate si fossero attivate le assunzioni previste per l'Arma dei carabinieri si sarebbe risolto assai meglio il problema del controllo del territorio con personale appositamente addestrato, piuttosto che usare le poche unità dell'Esercito poi destinate, uomini e donne che hanno peraltro anche diversa professionalità. Prima di concludere il mio intervento vorrei fare un'ultima brevissima considerazione. Siamo nei giorni che celebrano il 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Il 3 dicembre, ad Oslo, il sottosegretario Scotti ha sottoscritto per il nostro Paese la Convenzione di Dublino per la messa al bando delle bombe a grappolo. Queste sono munizioni micidiali, che oltre alle conseguenze immediate in guerra, a medio e lungo termine risultano terribili soprattutto per le popolazioni civili, creando morti, menomazioni gravissime e l'impossibilità di utilizzare per il lavoro agricolo vaste aree di territori dove magari sarebbe essenziale riprendere la vita normale in modo che non ci sia la fame. Siamo dunque assai contenti che il nostro Paese sia stato protagonista prima a Dublino ed ora a Oslo, così come lo siamo stati in passato per l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Ottawa per la messa al bando delle mine antipersona. Si allarga infatti in questo modo l'impegno nel mondo per il disarmo umanitario. Spero che lavoreremo tutti insieme per una rapida ratifica della Convenzione, così come a maggio abbiamo insieme prodotto, qui al Senato, una mozione di sostegno alla nostra alla nostra presenza a Dublino per la messa al bando delle *cluster* *bomb*. Ora è però indispensabile che il Governo si adoperi per colmare il vuoto creato dall'annullamento degli stanziamenti dedicati a tali attività umanitarie e di cooperazione. L'azzeramento del fondo per lo sminamento umanitario, di cui non c'è traccia in finanziaria, e che di fatto vanifica la possibilità di essere conseguenti alle indicazioni previste dalle Convenzioni, va coerentemente superato accogliendo gli emendamenti proposti e dando così credibilità all'atto della firma

precisazioni, visto che chi mi ha preceduto ha voluto fare addirittura il suo testamento biologico. Parto da questo aspetto: io sono felice di vivere fino a quando avrò la possibilità di farlo e sono disponibile ad aiutare chiunque avesse desiderio, bisogno o necessità di continuare a vivere, perché la vita è un miracolo e perché è dal rispetto della vita che discende tutto il resto.

Ogni volta che si parla di criticità della società si fa riferimento alle donne che lavorano di meno, a quelle che guadagnano meno, eccetera. Noi donne - vivaddio! - siamo diverse dagli uomini ma siamo persone normali. Anzi, siamo forse qualcosa di più: non dimentichiamo che le donne

volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, struttura introdotta con la legge di bilancio 2008; vorrei dire che si tratta di una piccola rivoluzione in termini di

un contenuto normativo estremamente snello e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, «in via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, micro/settoriale e localistico».

Fatta questa importante sottolineatura, è mio compito relazionare sugli argomenti del disegno di legge finanziaria 2009 di competenza dell'11a Commissione, nella cui sede ho già illustrato ai colleghi senatori le parti salienti. L'articolo 1, comma 4, del disegno di legge finanziaria ha introdotto un principio importante: le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria sono ora destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati. È anzitutto una questione di sensibilità sociale che, in un momento di difficoltà per il Paese, richiama ai doveri di solidarietà espressi dalla Costituzione; penso che tutto questo alla sinistra dovrebbe piacere. altresì di una scelta economica espansiva, fatta per arginare la diminuzione della domanda interna e per agevolare il rilancio economico. Relativamente al contenuto dell'articolo 2, comma 36, in attesa dì una riforma complessiva, viene comunque incrementato da 450 a 600 milioni di euro lo stanziamento per la concessione e per la proroga degli ammortizzatori sociali ciò in deroga alla normativa ordinaria. Abbiamo visto quanto è stato fatto per gli ammortizzatori sociali, anche per alcuni casi straordinari su cui non mi dilungo perché vorrei essere sintetica. I commi 37 e 38 estendono, a cominciare dal prossimo anno, il trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità, con il limite con il limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a vantaggio dei lavoratori dipendenti delle società di gestione aeroportuale o da esse derivate. I commi dal 22 al 24 del medesimo articolo 2 determinano l'adeguamento, per l'anno 2009, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche

(ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. Mi sembra dunque che si stia cercando di intervenire e di venire incontro di intervenire e di venire incontro a varie parti della società. Il comma 25, in conseguenza degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, prevede un riordino dei trasferimenti per le prestazioni previdenziali, disponendo, più specificamente, che non sono più a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l'INPS

inferiore a decorrere dal 2009, ossia 1.800 milioni di euro. I commi dal 27 al 31 recano ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. In esso leggiamo alcune importanti novità per far fronte alla congiuntura sfavorevole, ma soprattutto per evitare il prolungarsi delle trattative per i rinnovi dei contratti di lavoro. Ricordo che in molte occasioni si è arrivati alla firma degli accordi quando si era già prossimi alla scadenza ulteriore, con un acuirsi di tensioni, dannoso prima di tutto per i dipendenti oltre che per il buon funzionamento dei servizi pubblici.

ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico. Questo è molto importante perché, in aggiunta a quello previsto dall'articolo 3,